Signor Presidente, le agenzie di stampa stanno battendo in continuazione notizie di sempre nuovi incendi. L'Ufficio statistico ci dice che ieri è stata la giornata di maggiore siccità degli ultimi dieci anni. dieci anni. Anche nelle ultime ore l'emergenza della Sicilia e del Vesuvio ci dà il quadro di una situazione ancora più pericolosa. Mi sembra ci siano tutti gli estremi per chiedere che il Governo venga a riferire su quella che, minuto dopo minuto, sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Senatore Quagliariello, approfittiamo della fortunata presenza del ministro dei rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro, che farà da tramite per potere organizzare questa informativa.

nel Paese delle sempiterne emergenze da gestire con leggi che non risolvono nulla, anche questo decreto rientra nella diffusa modalità dei rappezzi.

Io sono favorevole alle vaccinazioni, che hanno permesso in passato e permettono oggi, di eliminare malattie infettive mortali e invalidanti come ad esempio la poliomelite. Nessuno qui sta mettendo in dubbio l'efficacia del metodo vaccinale. Oggi è la Ministra della sanità a chiederci, con toni fortemente allarmistici, una maggiore copertura vaccinale e per ottenerla ricorre a un allarmismo colpevolizzante per legittimare l'imposizione, l'autoritarismo e il timore di incorrere in sanzioni pesantissime. Non voglio, in questo mio breve intervento, affrontare il discorso dal punto di vista scientifico - non sono un medico - ma dati scientifici vengono branditi come armi in questa, a mio parere, vera e propria crociata sostenuta dalla Ministra e non voglio scendere allo scontro di dati contro dati. Analizzare i dati scientifici è comunque fondamentale, utilizzarli, però, in maniera strumentale come arma per la propaganda, da una parte o dall'altra, dove vince chi ha più violenza verbale o capacità di seduzione delle coscienze o influenza sui mezzi di comunicazione, conduce a una parossistica confusione e sfiducia delle famiglie nel sistema sanitario e nelle istituzioni. Capire perché vi è certamente un aumento della cosiddetta esitazione vaccinale in Italia, come dimostrato da studi molto accurati in Veneto e in Emilia-Romagna...

Non voglio, in questo mio breve intervento, affrontare il discorso dal punto di vista scientifico - non sono un medico - ma dati scientifici vengono branditi come armi in questa, a mio parere, vera e propria crociata sostenuta dalla Ministra e non voglio scendere allo scontro di dati contro dati. Analizzare i dati scientifici è comunque fondamentale, utilizzarli, però, in maniera strumentale come arma per la propaganda, da una parte o dall'altra, dove vince chi ha più violenza verbale o capacità di seduzione delle coscienze influenza sui mezzi di comunicazione, conduce a una parossistica confusione e sfiducia delle famiglie nel sistema sanitario e nelle istituzioni. Capire perché vi è certamente un aumento della cosiddetta esitazione vaccinale in Italia, come dimostrato da studi molto accurati sia in Veneto che in Emilia-Romagna, aiuterebbe la comprensione di cosa davvero la popolazione si aspetta da uno Stato regolatore, che in virtù delle leggi europee non controlla più nulla e non affianca davvero la popolazione su un tema di così vitale importanza. Terrorizzare e obbligare le famiglie, come fa questo decreto-legge, crea in definitiva solo maggior sospetto e allontanamento dalla profilassi vaccinale. A fronte di una minore copertura di gregge il Governo probabilmente non dice quali siano tutte le vere cause del problema. L'Italia in questi ultimi vent'anni ha conosciuto una forte presenza di popolazioni provenienti da diversi Paesi del mondo. La popolazione accolta è ormai superiore al 5 per cento dell'intera popolazione italiana. Ha potuto questa essere affiancata da medici di famiglia e da una sanità efficace? La popolazione caduta in stato di povertà è pari - ce lo dicono le statistiche - a più di 5 milioni di individui ed è in continua crescita. Siamo sicuri che le famiglie di questi individui possano pensare a informarsi e provvedere a vaccinare i propri bambini? La solidarietà è sacrosanta è intoccabile, ma questa è accompagnata da servizi pubblici efficaci e diffusi? Inoltre non si ha paura dei vaccini per la disinformazione, come ritengono i proponenti dell'obbligo vaccinale, ma è l'aria di sfiducia nel Sistema sanitario nazionale che aleggia tra i dubbiosi a dipingere una sanità che viene percepita dall'utenza come poco trasparente, poco dialogante e per niente attenta al paziente e questo purtroppo avviene in tante Regioni italiane. invece quanto sia fondamentale il rapporto di fiducia medico-paziente per l'efficacia della terapia, come d'altronde sancito nel codice deontologico medico. In fatto di vaccinazioni, dato che si tratta di un'azione preventiva, tale sentore può avere effetti molto più incidenti sul comportamento e sull'allontanamento da tale prassi, soprattutto in un momento storico che si avvicina all'emergenza ma che ancora non lo è, in cui gli effetti gravi delle malattie per cui ci si vaccina, non sono ancora così diffusi. Tutti qui vogliamo che non si diffondano. Ma attraverso cosa? Attraverso un servizio sanitario che informi, educhi, affianchi il cittadino e lo rassicuri, aspirando a uno Stato che renda tutti noi parte della comunità italiana attraverso principi di correttezza, trasparenza e partecipazione alle scelte. I tagli alla sanità, la tecnocrazia manageriale che ha invaso il settore sanitario, l'abbandono della figura del medico di base, i tagli all'educazione scolastica in materia sanitaria, che questo decreto-legge prova a tamponare in virtù dei rappezzi, in modo risibile, sono tra i principali colpevoli della diminuzione della copertura vaccinale in Italia. Su questi settori il Governo dovrebbe intervenire. Ma non si può, perché il *fiscal compact*, i parametri di Maastricht e la Commissione Europea ci impediscono di gestire le nostre risorse pubbliche interne anche e soprattutto in ambito sanitario. La coercizione è un atto di chiusura del dialogo tra istituzioni e cittadini, specchio di uno Stato che riconosce di non avere le risorse e le capacità per prendere provvedimenti diffusi in direzione educativa e di promozione della salute, oltre a decretare il fallimento della comunicazione in medicina tra operatore e paziente nell'ambito delle vaccinazioni e della prevenzione. Già il mio collega, dottor Romani, nel suo intervento di stamattina ha ribadito l'importanza del rapporto di fiducia strettissimo per la validità e l'efficacia della cura tra medico e paziente. II clima di fiducia, in seno al quale nasce e si sviluppa il senso civico, prevede correttezza, sempre, anche quando la sincerità è difficile da mostrare e la cultura della prevenzione e il rispetto delle istituzioni è ciò che a tutti i cittadini dovrebbe permeare da uno Stato rispettoso, depositario di fiducia e attento ai cambiamenti sociali. E va sottolineato e ribadito con forza che la funzione educativa di promozione della fiducia e di tutela della salute pubblica non può essere in alcun modo delegata a uno strumento quale la rete di Internet. Per la salute dobbiamo affidarci alla scienza, ma la scienza e lo Stato democratico affiancano, educano e non impongono. Questo decreto-legge dimostra nel modo più chiaro ed evidente che il Governo oggi non è in grado di assicurare tutto questo. *(La

per questo intervento mi è venuto in mente un libro che ho letto tanto tempo fa, scritto da un biologo e ottimo divulgatore scientifico che si chiama Jared Diamond, che ha scritto: «Armi, acciaio e malattie». Ciò che mi colpì fu il fatto che le malattie hanno decimato intere popolazioni delle Americhe: furono più le malattie dovute ai germi portate dai *conquistadores* a uccidere le popolazioni americane che non

mi sembra, per certi versi, che si sia tornati indietro. La cosa che mi colpisce è che sembra difficilissimo far comprendere alle persone che dietro la decisione di prevenire

In realtà, noi dobbiamo far fronte a un problema di globalizzazione, in cui viaggi, spostamenti, migrazioni e povertà vanno a braccetto con le nostre malattie, quindi una campagna di prevenzione può solo proteggere i nostri figli. i nostri figli. Per quanto riguarda gli adiuvanti che si inseriscono nei vaccini, i sali di alluminio sono stati in parte sostituiti e ci sono altri tipi di adiuvanti, molto più efficaci e che non danno reazioni avverse o perlomeno sono molto limitate.

a un certo punto bisogna adottare delle soluzioni molto importanti per la prevenzione e quindi per tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili.

quando dovevo vaccinare i miei figli chiesi consiglio a mia madre, che chiaramente aveva un'esperienza diversa dalla mia. Per la pertosse era prevista una vaccinazione facoltativa e non obbligatoria, ma lei mi raccontò che quando era piccola passò mesi e mesi con questa tosse canina e mi

che famiglie informate sulla necessità di fare vaccinazioni, nonostante tutto, erano molto titubanti e non erano proprio convinte di procedere alle vaccinazioni; viceversa, quando l'esperimento è stato condotto su un gruppo di genitori a cui venivano mostrati gli effetti concreti di queste malattie (quindi del vaiolo, della poliomelite, eccetera), la percezione cambiava e l'aderenza alla vaccinazione è stata assolutamente

tratta di un argomento molto ostico e importante, ma è pur vero che abbiamo una eredità importante, quella di pensare ai nostri figli che saranno le generazioni future che dobbiamo tutelare; soprattutto dobbiamo tutelare i più deboli e non possiamo pensare che lo Stato decida qualcosa che

che ieri alla Camera è stato votato con la fiducia il decreto-legge n. 99 del 2017, cosiddetto decreto banche, regalando 17 miliardi di euro per sanare i conti di banche private; 17 miliardi che avrebbero potuto essere utilizzati per un anno di reddito di cittadinanza. Questo come *incipit*, per mostrare attenzione e avviare un dialogo costruttivo con la cittadinanza tutta, poiché anche il decreto-legge che discutiamo oggi ha avuto un *iter*, oserei dire, oserei dire, inadatto e offensivo per la cittadinanza tutta. Mi piace ricordare che nell'articolo 32 della nostra Costituzione si specifica come: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno» - e ripeto: nessuno - «può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La legge dunque, non può in alcun modo superare i limiti imposti dal rispetto di questo. La Ministra ha spiegato che il provvedimento è stato scritto per tutelare i bambini, benché l'obbligatorietà, senza un serio e puntuale *iter* informativo, per il tramite di una rete di medici e pediatri che aiutino i genitori alla conoscenza del percorso vaccinale vero e proprio, viene definita per me "coercizione". Siete passati da un'obbligatorietà di dodici vaccini a una di dieci, ma con ulteriori quattro vaccini consigliati. Quindi abbiamo dieci più quattro. Ministro, questa vostra scelta di imposizione costringe le persone a soccombere a una legge, sull'indicazione positiva del termine «di tutela della salute pubblica», ma con incolmabili

andiamo con ordine, poiché nell'analisi degli articoli che in particolare vedono coinvolti gli istituti scolastici e il personale docente, all'interno degli articoli 3, 4 e 5, viene specificata la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi,

prevedendo che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero il termine del 10 settembre è assolutamente incongruo, visto che numerose scuole hanno date d'iscrizione È assurdo poi come la responsabilità della vaccinazione obbligatoria ricada solo e soprattutto sulla responsabilità dei genitori e, a cascata, dei docenti e dei dirigenti. Non ci si è posto minimamente il dubbio che questa responsabilità non ha senso che ricada su

2017-2018. E con quali finanziamenti? Sempre tramite il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Ecco che si prevedono ulteriori tagli alla didattica; meglio mantenere tutti ignoranti. Vi è poi il vergognoso emendamento che propone di consentire al Ministero della salute di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni (tra questi ci sono anche i sono anche i talassemici). Questo taglio ulteriore alla sanità pubblica è una vergogna, anche perché noi sappiamo in che condizioni sono gli ospedali pubblici di tutta Italia.

usando un discutibile metodo che crea dubbi, paure, confusione, ritardi nella realizzazione e migliaia di ricorsi che intaseranno la giustizia, da cui ci potremo sicuramente aspettare sentenze variopinte. Sappiamo già come mai in Italia dal 2012 ci sia stato un calo vaccinale: è stato grazie all'inchiesta della procura di Trani, che ha messo in relazione l'autismo con le vaccinazioni, relazione smentita da tutto il mondo scientifico internazionale. L'inchiesta si è conclusa dopo quattro anni affermando finalmente che non c'è nessun nesso non c'è nessun nesso tra l'autismo e le vaccinazioni, ma ormai il danno era fatto, infatti c'è stato un calo notevole di vaccinazioni, soprattutto in Puglia. Negli anni successivi al 2012 non c'è stato un sufficiente monitoraggio, eppure c'era già l'obbligo vaccinale con sanzione, ma solo dieci ASL hanno fatto segnalazione nel 2016. Non c'è stata in questi anni una campagna informativa seria, non risibile come quella attuale, che avrebbe dovuto precedere il decreto-legge. Invece anche ora l'informazione è fatta male anche da chi dovrebbe per conoscenze scientifiche, difendere il principio dell'importanza del valore delle vaccinazioni. Mi riferisco ad esempio a un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; mi riferisco a una trasmissione televisiva su La7, seguita da milioni di persone,

Tutti abbiamo salutato con grande condivisione un piano vaccinale perfetto, messo a punto dal Ministro della salute, ove si dava grande rilievo alla formazione e all'informazione, ma questo piano è stato praticamente annullato dal decreto-legge stesso. Durante le audizioni in Commissione sanità, abbiamo avuto esperti dell'Associazione dei pediatri, abbiamo ascoltato Garattini dell'Istituto Mario Negri, la dottoressa Salmaso tutti hanno espresso dubbi e criticità sul metodo. Abbiamo udito i rappresentanti delle Regioni come Saitta e direttori delle ASL, e tutti hanno espresso dubbi e difficoltà

Sappiamo che il calo delle vaccinazioni, oltre alla magistratura, è dovuta a *talk show* in cui parlano opinionisti che non hanno una minima base scientifica e, purtroppo, anche l'ordine dei medici si è svegliato un po' tardi. tardi. Anche i medici di famiglia e i pediatri di famiglia non si sono spesi abbastanza in questi anni, a meno che non avessero dati per sapere che c'era un calo delle vaccinazioni.

leciti. Ha dato modo a un popolo, al micropopolo no vax di avere argomenti per mettere dubbi a genitori allarmati per la violenza legislativa che ha fatto supporre le peggiori cose, compresi i conflitti di interesse. Presidente, io faccio parte di una generazione che ha avuto a scuola compagni con la poliomelite. Faccio parte della generazione i cui genitori, quando c'era una febbre alta, tremavano, perché magari i figli di amici erano morti per la difterite o la pertosse, credo che vaccinare i propri figli sia un grande gesto d'amore e responsabilità per il loro bene ed è più importante delle ansie che qualsiasi genitore può avere prima della loro vaccinazione. Non condivido la scelta di alcuni, per ideologia, di non far vaccinare i propri figli, sfruttando anche quell'immunità di gregge, per preservarli comunque dalle malattie, sfruttando i benefici delle ansie di altri che decidono di vaccinare i propri figli per senso di responsabilità.

Signor Presidente, ringrazio i colleghi, senatrici e i senatori, quelli che sono intervenuti e quelli che ringrazio la relatrice, non solo per il ruolo attento e responsabile che ha svolto nei lavori di Commissione, ma anche per la sua relazione all'Assemblea, assolutamente conforme - nello spirito e nella lettera - al dibattito che ha investito diversi profili della materia vaccinazioni. Ne tratterò alcuni, quelli che, a mio giudizio, ritengo più attinenti al merito del provvedimento e soprattutto qualificanti le scelte che hanno guidato e motivato le proposte di emendamenti approvati dalla Commissione. Il primo profilo attiene al rapporto tra impianto tecnicoscientifico del provvedimento e potere legislativo, una fattispecie particolare di un tema molto più grande che affronta i rapporti tra scienza e politica. La sottile linea di confine che separa l'autonomia della scienza e il potere legislativo è stata, è e sarà oggetto di riflessioni e ricerche che abbracciano più discipline del sapere umano: la filosofia, l'antropologia, l'etica, la bioetica, la storia della medicina, l'epistemologia, il diritto, il biodiritto e il diritto costituzionale. Sul piano concreto, nell'esercizio del potere legislativo, è proprio la giurisprudenza costituzionale a indicare la strada e, tra le tante sentenze in materia, vi leggo un passaggio della sentenza n. 282 del 2002, che considero la più vicina alle nostre fattispecie.

«Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali» - è un inciso che nella fattispecie riguarda i trattamenti sanitari obbligatori «non é, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione». Si tratta di una sentenza, che, peraltro, contrastava con una legge regionale che intendeva abolire una pratica - diciamo diciamo così - incivile nel trattamento di alcuni disturbi psichiatrici, oltre che inappropriata. Dunque, i fondamenti tecnico-scientifici su cui poggiano le proposte vaccinali hanno una loro autonomia dall'azione del legislatore. Il razionale della loro indicazione, somministrazione e valutazione degli esiti è tutto all'interno del metodo scientifico, quello che dagli inizi del 1800 ha profondamente trasformato le scienze naturali, compresa la medicina, che così è diventata scientifica. Il metodo scientifico applicato alla medicina ci consegna in questa fase storica della sua evoluzione le evidenze di varia forza; indirizza la ricerca e la sperimentazione sui principi di ripetibilità delle prove - cito in questo senso la falsificazione di Popper - che valuta gli esiti dei trattamenti sulla base del rigore dei *trial*, delle meta analisi e così via. Nel concreto del nostro provvedimento, la rimodulazione degli obblighi vaccinali proposti dalla Commissione rispetta quel limite tra scienza e politica, perché non incide sulla struttura tecnico-scientifica del provvedimento, ma, nel riconfermare la rilevante necessità di proteggere e prevenire da malattie con vaccini sicuri ed efficaci - quelli presenti nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale prefigura solo una diversa strategia operativa, peraltro condizionata nel tempo, per conseguire quegli obiettivi e non altri. Al riguardo, ho molto apprezzato il taglio di alcuni interventi, prevalentemente strutturati sull'architettura tecnico-scientifica del provvedimento;

Al di là delle conclusioni assunte, alcune delle quali non sono da me condivise - ricordo che, anche nel maneggiare dati della letteratura scientifica, valgono alcune regole, quelle proprie del metodo scientifico in ogni caso sappiamo tutti e dobbiamo esserne consapevoli che le evidenze non sono verità assolute. La misura degli esiti non ha indicatori assoluti. La complessità e la variabilità biologica di ogni forma vivente, compreso l'uomo, rendono mutevoli o meglio evolutive le risposte ai trattamenti. Innanzitutto, non sono l'affollamento di pubblicazioni su «PubMed» o la citazione di singoli lavori che possono fondare affermazioni scientifiche impegnative. In tanto disordine si corre il rischio che ciascuno possa prendere dagli scaffali quello che ritiene più utile. Lo abbiamo già visto: il metodo Stamina era fondato su due pubblicazioni - credo - della Bielorussia. Ma soprattutto bandirei da questa discussione l'espressione «sperimentazione di massa», per due ragioni. La prima è assolutamente tecnica:

che sono stati sottoposti alle vaccinazioni, alla gran parte delle vaccinazioni oggi ricompresa nella fascia obbligatoria. La seconda ragione è che questa è un'espressione retorica - diciamo così che non aiuta il dialogo, che lo radicalizza e che, soprattutto, ricorda pratiche e culture totalmente estranee al nostro Paese e ai valori costituzionali di rispetto della libertà e della dignità dell'essere umano, dal codice di Norimberga, passando per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fino alla Convenzione di Oviedo e alle regole assolutamente trasparenti che governano la sperimentazione sull'uomo, e non solo sull'uomo, nel nostro Paese. Altri profili, invece, sono di stretta competenza del legislatore. Mi riferisco a quella domanda forte e corale di informazione, di trasparenza, di rassicurazione sul controllo dei rischi connessi alle pratiche vaccinali. Dalle audizioni, dai dialoghi, dai confronti sono emersi ritardi delle organizzazioni sanitarie a dotarsi di strumenti di governo delle politiche vaccinali. Sono poche le Regioni che possono vantare anagrafi vaccinali adeguate e soprattutto interagenti. È con questo provvedimento che viene finalmente prevista un'anagrafe vaccinale nazionale. nazionale. Dobbiamo dire - e da questo punto di vista inviterei il Governo a metterlo in agenda - che il duro contenimento del finanziamento della sanità in questi anni è passato anche per i centri vaccinali. È passato anche di lì: non erano vaccinati da questo. E ciò ha lasciato molti segni di sé: blocchi del *turnover*, precariato, scomposizione dei *team* multiprofessionali, che sono l'anima e l'essenza di un servizio di prossimità alle famiglie nella tutela della salute pubblica. Anche io - come già hanno fatto

altresì, l'evidenza che le posizioni no vax, ancorché aggressive sul piano mediatico e verso cui va tenuta alta la guardia, sono comunque l'epifenomeno estremo, radicale e minoritario di un fenomeno più vasto e carsico, che attraversa la medicina moderna e la moderna sanità. Può sembrare paradossale, ma anche la medicina delle evidenze può non essere autosufficiente quando deve calarsi nell'universo di ogni persona a cui si rivolge; quando deve confrontarsi con i valori di riferimento a cui ogni persona ispira il proprio vissuto; quando deve colmare la distanza con le paure; quando deve negare le false speranze che la disperazione sempre produce; quando deve indicare e rendere pubblici i propri limiti. Anche i vaccini, che tutta la comunità scientifica internazionale colloca tra i presidi di sanità pubblica dall'elevato indice costo-efficacia e sicurezza-efficacia, hanno bisogno di essere spiegati alle famiglie,

voluto leggervi qualche pezzo della lettera che ci ha inviato il direttore generale della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità

tutte quelle raccomandazioni assolutamente necessarie e urgenti e soprattutto funzionali a riorganizzare un moderno sistema nazionale nazionale di prevenzione vaccinale. È vero che esse erano presenti in un documento splendido e meraviglioso, come il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, ma qui le abbiamo trasferite

Sulle sanzioni avete già sentito che il lavoro è stato molto attento e sobrio: siamo stati davvero molto accorti e vedrete che lo saremo ancora in questa sede sul tema delle sanzioni. Rimane il problema dell'obbligo, che ho sentito essere contrario ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 32 della Costituzione.

l'istanza mossa da un pretore di Bassano del Grappa riguardante l'obbligo della vaccinazione anti-tetanica, anti-epatite B, anti-difterite

che il trattamento sia diretto non solo a migliorare e preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare la salute degli altri, perché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quell'autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto alla salute di ciascuno, in quanto diritto fondamentale. La seconda condizione

nella norma sono previste esenzioni connesse allo stato di salute e ricettività del soggetto, in modo che non determini danno. è che, nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto a trattamento obbligatorio, sia comunque prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato. A ciò potrebbe aggiungersi anche un risarcimento, qualora la condotta dei professionisti dei centri vaccinali non abbia rispettato le regole per colpa (articolo 2043 del codice civile). Nel provvedimento abbiamo chiaramente

abbiamo in carico. e assumere le libere determinazioni su questo tema, che - lo ricordo - è difficilissimo, perché attiene alla tutela della salute dell'individuo attiene alla tutela della salute dell'individuo anche in ragione dell'interesse collettivo. E questo aspetto è davvero molto complicato. Presidente, riavvolgiamo il nastro e torniamo col tempo a maggio. Cerchiamo di capire come avrebbe ragionato un padre di famiglia al posto del ministro Lorenzin. Non dico uno scienziato, non dico un medico e neanche un laureato, visto che il Ministro non lo è, ma la diligenza di un buon padre di famiglia -questa sì - me l'aspetto da un Ministro. È un criterio sancito anche dalla Cassazione. Torniamo dunque al mese di maggio di quest'anno. Abbiamo un'epidemia? Un nuovo virus dall'Africa? Il Ministro della salute in questo caso mette in campo ogni misura per fronteggiarlo. Ma non è questo il caso. Abbiamo scoperto una grave carenza all'ultimo momento, creatasi magicamente e immediatamente nella copertura vaccinale? Neanche. Per alcune malattie siamo di pochissimo sotto il tasso di vaccinazione ideale; per morbillo, rosolia e parotite siamo all'86 per cento circa: non distanti da altri Paesi europei, peraltro.

Lo dice Endrizzi? No. Lo dice il piano vaccini di gennaio e lo riconosce anche il presidente del Consiglio Gentiloni. Ma cosa abbiamo dunque? Abbiamo un aumento dei casi sull'anno precedente che non va trascurato. Per tutte le malattie? No, per il morbillo. Ora, questa è una malattia che ha fluttuazioni annuali. Nel 2008, con un tasso di vaccinazione superiore a quello attuale, furono comunque 5.312 i casi. E non lo dico io, ma EpiCentro, il portale epidemiologico del Ministero della salute. caso, un buon padre di famiglia, per il principio di precauzione, si pone il problema e si chiede: che obiettivo voglio raggiungere? La migliore copertura vaccinale. Diciamo che vorremmo superare il 95 per cento, soglia indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità. E come ci arriviamo? Un padre padrone

e si fa come dice lui. Con quali esiti poi è da vedersi perché, se con gli obblighi si ottenesse la *compliance*, si ottenesse la *compliance*, allora tutti pagherebbero le tasse. Ma sappiamo che non è così, perché è importante far capire i cittadini. I cittadini pagarono volentieri una tassa, e la pagarono volentieri perché fu spiegata. Parlo della tassa per entrare nell'euro, anche se poi quell'euro ci ha traditi. I cittadini pagarono volentieri quella tassa. E oggi, se venisse spiegata in termini scientifici e in un rapporto diretto tra il medico e la famiglia l'importanza del vaccino, non avrebbe paura di essere indimostrabile. sarebbe questo il requisito principale. Allora, un buon padre di famiglia non adotta lo strumento del decreto-legge, peraltro incostituzionale perché non ci sono un'emergenza, una necessità o un fatto eclatante comparso immediatamente e improvvisamente; un fatto, peraltro, che va in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione disponendo un trattamento obbligatorio. Non è possibile. Quando anche si tratti di contemperare il diritto alla salute della collettività e del singolo, è comunque necessario mettere in campo degli accorgimenti, ad esempio - verificare le possibili complicanze e informare i cittadini sulle possibili conseguenze, lasciando comunque una responsabilità e un margine di arbitrio. È quello che definiamo il consenso informato, che è un principio cardine della medicina che trova le sue radici negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ripreso poi dalla Convenzione di Oviedo, ratificata dall'Italia, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Governo ci ha sbandierato non meglio precisati impegni europei. È una falsità. Un padre di famiglia si informa e verifica dove, in Europa, abbiamo i migliori tassi vaccinali e le migliori pratiche. E si scopre che queste coincidono con i Paesi in cui non vige l'obbligatorietà: Francia, Germania e Inghilterra. In Francia - come ho già detto - sono tre i vaccini obbligatori, mentre in Inghilterra e Germania zero. Come arrivano allora a questi risultati? Attraverso l'educazione, ha detto prima la collega Rizzotti,

i figli della sua Nazione a rinunciare alla scuola, laddove peraltro la Costituzione prevede l'obbligo di istruzione. Un padre di famiglia non dispone sanzioni che consentono alle famiglie ricche di sottrarsi a un obbligo e non dà alcuna Non consente a chi ha gli strumenti economici per garantire comunque l'istruzione parentale ai figli, attraverso istitutori privati,

interagire le diverse anime, le sensibilità e il proprio elettorato di riferimento, e non in un decreto-legge che porta le ragioni, forse elettoralistiche, di una maggioranza sempre più scassata e allo sbando. Questa è la via.

del rapporto tra Parlamento e Governo e anche della voce dei cittadini che hanno il diritto di vedere rappresentata qui dentro. Siamo di fronte a un atto unilaterale che isola sempre più Governo e maggioranza in una torre d'avorio relega il buonsenso fuori da quest'Aula. È molto facile agitare strumenti e argomenti come questo, dove si radicalizza lo scontro tra posizioni

svilisce il senso di cittadinanza, il senso di coesione del Paese e porta a fratture e a imbarbarimento. Questo state proponendo, anzi state imponendo. Presidente, quando abbiamo anche la prova provata dell'incongruenza interna degli assunti del Governo, perché prima impone dodici vaccini e poi si accorge che dodici vaccini obbligatori non li ha nessuno e allora ne toglie due - così siamo almeno pari alla Romania

Forse, gratta gratta, scopriremo veramente che non c'è bisogno di dieci vaccini obbligatori, anche perché l'esempio del Veneto ci dice che il tasso vaccinale è molto buono, anche se può essere migliorato, senza che vi sia quell'obbligatorietà. queste ipocrisie, svelate anche nel recente passaggio in Commissione,

ampio e approfondito. Riprenderò alcuni dei punti principali della discussione che rientrano nel provvedimento e che sono stati anche oggetto interessante di confronto. Parto dalla modifica del comma 1 dell'articolo 1, e cioè della rimodulazione dell'obbligo, che è stata appena ripresa in modo approfondito dal senatore Bianco nel suo precedente intervento

poi declinato l'obbligo in tre livelli diversi: un'obbligatorietà che fa riferimento ai vaccini storici, un'obbligatorietà dettata dall'emergenza e un rafforzamento della raccomandazione. Sul rafforzamento della raccomandazione voglio rassicurare il senatore Aiello che, nel suo intervento, ci ha richiamati a non sottovalutare e i rischi della meningite che la vaccinazione anti-meningococco B e C può invece risolvere. I vaccini raccomandati, come tutto il Piano nazionale vaccinale,

È soprattutto la cadenza triennale cui è sottoposto il secondo blocco di vaccini che lascia aperta l'opportunità di riavere all'interno anche delle Camere una relazione motivata da parte del Governo sull'eventuale scelta di rinnovare l'obbligo o di rimodularlo, che permetterà di seguire e far convivere i due strumenti dell'obbligatorietà e della promozione attiva in modo sussidiario, al fine di poter fare prossimamente prevalere e mantenere la promozione attiva. Sarà anche quella l'occasione - secondo me - nelle prossime cadenze triennali, quando un sistema vaccinale potrà definirsi più robusto e maturo, per affrontare i temi dell'esitazione vaccinale, ripresi da più senatori - ricordo quello della senatrice Dirindin perché è effettivamente una richiesta che esiste, ma che probabilmente in questo momento difficilmente riesce a convivere con una situazione di emergenza.

Un secondo punto che il dibattito ha affrontato concerne la difficile ricerca di un equilibrio tra libertà personali e salvaguardia della salute collettiva. Ha ragione il senatore Romano nel ricordarci che la salute non è solo un diritto primario dell'individuo, ma anche un interesse preminente della collettività. Sul valore sociale delle vaccinazioni, senatrice Puglisi, abbiamo riflettuto tutti insieme. è stato anche ricordato quanto, nell'affrontare questo dibattito, ognuno di noi, ognuno dei partecipanti al dibattito anche esterno, porta il proprio bagaglio di storia e di cultura. senatrice Maturani e il senatore Buemi hanno ricordato un periodo storico in cui il timore della poliomelite era così pesante da essere un macigno sulle spalle dei genitori e di come allora si vide con sollievo l'arrivo di uno strumento per contrastarla sia per garantire salute, sia soprattutto per guardare con serenità al futuro dei propri figli.

il dato sull'obbligatorietà o sulla somministrazione di vaccini nei Paesi europei. Dovrebbe essere un dato quasi trasparente, ma abbiamo sentito termini diversi. utilizzare notizie non precise o condivise aiuta a diffondere la disinformazione. Proprio su questo tema, anche in sede di elaborazione del disegno di legge di conversione, abbiamo voluto insistere, lavorare

che c'è bisogno che le informazioni sugli eventi avversi non siano una leggenda o una favola, ma siano sancite, stabilite, pubblicate e rese sicure anche nella loro lettura.

singolo per avere contezza del proprio stato vaccinale nel tempo e per poter utilizzare quella fase su cui abbiamo molto lavorato e anche molto insistito, la dovuta, necessaria semplificazione burocratica all'interno del sistema scolastico, al fine di agevolare le famiglie, ma anche gli uffici delle aziende sanitarie e delle scuole, in un trasferimento di dati che a un certo punto dovrà essere pubblico, noto e condiviso, senza creare un giro di certificati non più all'altezza dei tempi.

Abbiamo analizzato questo aspetto e abbiamo riscontrato in tanti che proprio una delle cause della riduzione delle coperture vaccinali è dovuta alle conseguenze dei tagli che i sistemi territoriali e i servizi vaccinali hanno subito come peso. È stato fatto tanto lavoro. La Commissione ha lavorato molto e ha audito tutti. Lo dico perché voglio fare un'osservazione rispetto all'intervento del senatore D'Anna,

Tutti coloro che hanno potuto partecipare ai lavori della Commissione igiene e sanità, pur convinti oppure in forte contrapposizione, hanno potuto constatare quanto invece sia stato approfondito e anche faticoso, ma puntuale, il lavoro svolto; e di questo

all'avvicinarsi alla vaccinazione, voglio anche sperare che la discussione di questi giorni e delle ultime ore possa lanciare al Governo e al Ministro un segnale forte dell'importanza della vaccinazione e soprattutto farli guardare al futuro, al campo della ricerca, alla creazione di nuovi vaccini e a una sempre nuova e migliore loro produzione. E lo dico lo dico perché la ricerca deve essere continua e costante e questa deve essere la sua evoluzione. É evidente che l'innovazione, anche con nuovi metodi di somministrazione, può facilitare un'avversione all'utilizzo di ago e siringa - è uno dei fattori - perché esistono malattie antiche, come la tubercolosi e la malaria, rispetto alle quali è necessario trovare ancora delle soluzioni, così come vi di nuove epidemie (ricordo Zika ed Ebola) che diventano sempre momento di paura quando le notizie arrivano attraverso i giornali. Non ultime, le sperimentazioni oppure le opportunità, che possiamo vedere, di avere dei vaccini anche contro alcune forme tumorali. L'invito è, quindi, di rafforzare l'investimento sulla ricerca e sulla produzione di vaccini, per una salute futura sempre più tutelata. più tutelata. Come un gatto che si morde la coda, si può pensare di tornare al punto uno. Nel momento in cui si parla di nuove produzioni di vaccini e di nuova ricerca, dobbiamo pensare, avendo una responsabilità non solo locale e non solo nazionale, con uno sguardo più ampio, alla necessità di produrre e fornire vaccini anche a quei Paesi e a quelle popolazioni che oggi non ne hanno la massima fruizione. Là dove si muore, dove i bambini muoiono, si vorrebbero avere medicinali per salvare se stessi e i propri piccoli. Noi, che per fortuna viviamo un momento di maggiore benessere, dobbiamo invece affrontare il dubbio e la paura. Per le famiglie i timori e le paure sono più che comprensibili. Noi, invece, abbiamo la responsabilità di dare loro delle risposte, di evitare le strumentalizzazioni e di pensare

gentili senatrici e gentili senatori, desidero innanzitutto esprimere il mio più vivo ringraziamento per il dibattito che si è svolto in modo veramente costruttivo in Commissione. Vorrei ringraziare i tecnici

l'obiettivo che credo tutti noi ci stiamo dando, anche coloro che possono avere delle posizioni in quest'Aula, e cioè di garantire la sicurezza della nostra collettività. Il percorso del lavoro in Commissione non è stato semplice, ma è stato complicato. Ma, come ho sempre detto, io ho un atteggiamento estremamente laico di fronte a questo tema, e poi vi dimostrerò perché. Secondo me, non si tratta di una questione di appartenenza politica, non riguarda l'essere membri di un partito o di un altro, stiamo affrontando uno dei temi più grandi e più importanti di sanità pubblica: quello delle profilassi vaccinali, della copertura e dell'immunizzazione della nostra società. È un tema estremamente importante e solo chi

nuovamente casi di pertosse nei reparti neonatali dopo vent'anni che non li vedevano più, e chi si è ritrovato nei nostri grandi ospedali nel Lazio, in Veneto, in Sicilia, in Lombardia, in Campania, per citare solo alcune

Oppure le tante persone ammalate, affette da una patologia...

Io credo una cosa, signori. Stiamo parlando della vaccinazione del Paese; stiamo parlando dell'immunizzazione dei nostri figli e credo che sia interesse di tutti ascoltare le ragioni del Governo e ascoltare le ragioni, visto che sono state sollecitate da più parti, che hanno spinto il Ministro della salute a prendere questo provvedimento. Possiamo farlo in quest'Aula o sui giornali. *(Commenti della senatrice De Pin)*. Credo che quest'Aula rispecchi il senso dell'istituzione che tutti i senatori rappresentano qui UPT)-PSI-MAIE))*, in cui si rappresentano 60 milioni di italiani. Stiamo parlando di una questione che riguarda la salute di tutti. salute*. Anche delle persone che ancora devono nascere, quindi di coloro che nasceranno nei prossimi anni, e speriamo in modo sempre maggiore. Quest'anno le vaccinazioni hanno salvato nel mondo 2.500.000 vite.

che danno l'idea dell'importanza delle vaccinazioni. Mentre noi stiamo facendo qui questa discussione, dall'altra parte del mare, dall'altra parte del mare, del nostro Mar Mediterraneo, i Paesi ci chiedono di aiutarli a vaccinare i loro figli, per queste vaccinazioni che noi rendiamo obbligatorie. Questo non perché abbiano esitazioni vaccinali, ma perché non hanno le risorse economiche per acquistare e garantire questi vaccini che salvano la vita ai loro figli e alle persone adulte. Permettetemi, però, di fare un passo indietro e di raccontare qui come siamo arrivati alla proposizione di questo decreto-legge.

della copertura delle vaccinazioni in Italia. Durante il dibattito, molti si sono chiesti come sia possibile che il Governo non si sia accorto prima che eravamo caduti nell'immunizzazione di massa; che, mano a mano, negli anni, abbiamo avuto un calo della copertura vaccinale nel nostro Paese. Sì che ce ne siamo accorti.

abbiamo sensibilizzato le Regioni a campagne vaccinali; abbiamo cominciato a parlare sempre più di vaccinazione, dell'importanza della vaccinazione e del fatto che non esiste alcuna correlazione scientifica tra vaccinazione del morbillo e insorgenza dell'autismo. Nessuna. Sì, perché questo è uno dei fattori che hanno scatenato questa specie di postverità; parlare di *fake news* è troppo nobile: una menzogna che ha avvelenato i pozzi della cultura scientifica e sanitaria di intere popolazioni. Abbiamo cominciato a lavorarci. Abbiamo predisposto un Piano nazionale vaccini

gli indici, l'insorgenza dell'epidemia di morbillo hanno dimostrato come abbiamo necessità in questo Paese di recuperare intere coorti di bambini non vaccinati che si sono sommate anno per anno. Il problema non è certo l'87 per cento di bambini vaccinati contro il morbillo a fronte di un 95 per cento di quest'anno, ma quanti bambini abbiamo perso negli ultimi dieci anni: 50.000, 60.000, 70.000 l'anno, moltiplicati per decenni. Questo ha comportato il fatto che nel nostro Paese abbiamo dei buchi, e quello che vediamo nelle statistiche dei dati, queste cifre (92, 87, 85)

parlando ai propri cittadini e alle proprie classi dirigenti, dicendo: abbiamo un'urgenza, che non è semplicemente programmatoria, da qui a dieci anni. L'urgenza è far salire questo basso livello di immunizzazione in modo veloce, rapido; cioè, in sicurezza la collettività. Questo è il senso dell'articolo 32 della Costituzione, che sancisce non solo il diritto alla salute individuale, ma il dovere dello Stato di garantire la salute collettiva, la sicurezza collettiva in un sistema universalistico come il È per questo che siamo intervenuti con l'obiettivo di far risalire in modo veloce le coperture vaccinali. ho ascoltato moltissime indicazioni, ma ci sono momenti in cui, a proposito del buon padre di famiglia, anzi, parliamo della buona mamma di famiglia, visto che sono le donne che prendono queste decisioni nelle nostre famiglie,

prevenzione e che salvano la vita dei nostri figli; che non vogliamo averesulla coscienza le persone negli ospedalie che abbiamo interesse alla sicurezzacollettiva*.

salute*. Ho sentito molte cose in quest'Aula e spero veramente che vi sia un invito alla ragionevolezza nel prosieguo del dibattito.

senza interruzioni. Non mi costringete a prendere provvedimenti che non voglio prendere. Prego, concluda, signor Ministro.

che dice che le strategie di vaccinazione legate all'iscrizione scolastica hanno dimostrato di essere efficaci in molti Paesi per evitare epidemie nelle scuole e ottenere un'alta copertura vaccinale. Continua citando i casi, ad esempio quello della California, dove questo è stato fatto proprio per il morbillo, portando l'obbligatorietà a nove vaccinazioni

di tutta la comunità medica italiana, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e di quelli ospedalieri, dei consultori familiari, di tutte quelle figure che sono accanto alle madri e ai padri

più parlare di bambini che sono morti o di persone adulte che si trovano in condizione gravi, per malattie che possono essere semplicemente evitate con una vaccinazione,

sulle complicanze o sulle nanoparticelle, temi su cui avremo sicuramente modo di entrare approfonditamente nel merito durante la discussione degli emendamenti: vale la pena di farlo, per tranquillizzare le persone e per istituire anche un dibattito sulla verità scientifica, sulle tante cose che ascoltiamo e che vengono dette e ripetute, spesso - anzi, direi sempre - senza alcuna evidenza. Fatemi però fare un richiamo al ruolo di questa

Abbiamo ingaggiato un dibattito durato più di un anno e molte delle questioni che sono state sollevate le abbiamo qui risentite. un dibattito che ha portato alla luce la verità vera e provata e la non verità che c'era dietro. Questa Assemblea ha vinto

Siamo alla fine della legislatura e siamo di nuovo di fronte ad un dibattito sull'antiscienza. Questo è il segno del nostro tempo, ma è anche il segno della grande responsabilità che tutti i membri di questa Assemblea hanno - non per oggi, ma per i posteri e che questo Ministro ha di fronte al Paese. È una responsabilità che viene prima di tutto ed è quella di affermare la verità dell'evidenza scientifica a fronte delle post-verità di porsi come baluardo per la sicurezza collettiva e la salvaguardia del nostro Servizio sanitario nazionale. Sono misure come questa che ci permettono di avere ancora un sistema universalistico considerato tra i migliori al mondo e di avere i nostri medici e i nostri ricercatori, che sono tra i più qualificati Quindi, quando i nostri ricercatori e le nostre istituzioni scientifiche parlano, parlano persone e istituzioni con grande autorevolezza e la politica, di fronte alle istituzioni scientifiche, deve fare un passo laterale *(Applausi dai non determina la scienza. La politica, se è buona politica, accompagna le scelte scientifiche, le spiega, le gestisce, le regola della senatrice Montevecchi)*, perché siamo qui, insieme, a batterci per garantire l'accesso dei nostri cittadini, non solo alle terapie innovative, ma anche a quelle che sono *old style*, ma che permettono a tutti di vivere in salute e in sicurezza.

si è voluto creare un dibattito falso, in cui si vuole evidenziare una presunta contrapposizione tra chi è favorevole ai vaccini e chi è contrario, ma non è questo il dibattito

di multe e di un rapporto conflittuale con i cittadini è uno strumento utile ad aumentare il livello di vaccinazione e di convinzione delle famiglie che le vaccinazioni siano utili o è uno strumento che mina questo rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. *(Commenti del senatore abbiamo le idee chiare, perché il Ministero della salute ha autorizzato la Regione Veneto ad attuare una politica diversa rispetto a quella dell'obbligatorietà, che è fatta di comunicazione, informazione e rapporto continuo e costante con le associazioni free vax per cercare di spiegare qual è l'utilità delle politiche delle vaccinazioni. Questo modello ha funzionato e continua a funzionare. E voi volete distruggerlo utilizzando un meccanismo totalmente diverso, basato su un atto di forza e di arroganza contro la libertà di scelta delle famiglie, e un atto di irresponsabilità politica, perché non

In nessuna parte del mondo esiste la possibilità per il Governo di utilizzare la forza, la coercizione e la punizione e la punizione per superare una forza che è ancora maggiore, cioè la volontà delle famiglie di tutelare la salute dei propri figli. Voi avreste dovuto convincere le famiglie dell'utilità delle politiche delle vaccinazioni e perseguire quella politica che - ripeto - abbiamo

fare delle audizioni, si sono toccate delle punte così alte di conoscenza, della qual cosa però dubito, perché qua stiamo ponendo un problema semplice, a cui voi vi ostinate a non voler dare una risposta. E vi arrabbiate pure. Prove di microscopia elettronica fatte in diverse università, non solo italiane, hanno dimostrato che all'interno dei vaccini, tranne quello per immunizzare il gatto, la presenza di una serie di sostanze quali la plastica, il tungsteno, l'acciaio, l'alluminio, di tracce di metalli e, di recente, anche la presenza di qualche centinaio di nanogrammi di mercurio. mercurio. Rispetto a questa evidenza, qualcuno si preoccupa di chiedere dei vaccini puri, che non contengano queste fetenzie? C'è qualcuno che vuole rispondere, il Ministro, il Presidente della Commissione sanità, gli autorevoli e eminenti uomini di scienza, medici, farmacisti, chirurgi, a un povero biologo, a un mentecatto come me? me? Volete risponderci? Volete rassicurare le mamme che stanno là fuori, sotto il solleone, con i propri bambini, che non mi sembrano l'esercito di Valmy, e neanche mi sembrano delle Erinni che stanno qui a conculcare la vostra scienza? Sono delle persone che non vanno

Probabilmente, quella che lei chiama non scienza non è ancora una scienza appurata e certificata, come molte delle cose che la scienza ufficiale dice di avere certificato e che non ha certificato. Ci dovreste, infatti,

perché non è possibile aprirsi a un confronto con eminenti virologi e scienziati, con qualcuno che sa certamente qualcosa più di me,

Allora, signor Presidente, sia indulgente. Il Ministro ha citato l'articolo 32 della Costituzione. È vero, lo Stato deve provvedere, ma quando c'è una minaccia per la salute, non quando ci alziamo cervelloticamente e diventiamo l'unico Paese che l'Organizzazione mondiale della sanità individua come punto di riferimento delle campagne vaccinali. E balziamo in vetta alla classifica dei vaccini obbligatori, nel mentre Paesi sottosviluppati come l'Inghilterra,

Io non nutro certezze. Gli uomini di scienza non ne hanno. Credo che il Ministro dovrebbe leggere qualcosa sull'epistemiologia popperiana, sulla filosofia della scienza, sul fatto che nella scienza tutto viene valorizzato per le prove di falsificazione per la prova di ripetizione. Nei vaccini c'è la fetenzia che non deve esserci. Quei vaccini inoculati in bambini di tre o dodici mesi vanno a disturbare e a interferire con un apparato immunitario: su questo non ci sono dubbi. Allo stesso modo la scienza ufficiale ci dovrebbe spiegare da dove viene fuori l'aumento delle allergie, delle malattie autoimmuni e di determinate patologie cancerogene. Perché la scienza ufficiale è così incapace di dare risposte e quando altri scienziati formulano delle ipotesi

dei vaccini puri che non contengano queste sostanze. Questo è quello che stiamo chiedendo: che lo Stato non faccia il gradasso a dire: «O vi mangiate questa minestra «O vi mangiate questa minestra o vi cacciamo dalla finestra». Voglio dire un'ultima cosa per non disturbare gli amici che vivono di certezze e che stanno dall'altra parte dell'emiciclo. Vedo il senatore Mirabelli molto nervoso e non voglio disturbarlo.

Romani, come da qui a poco vedremo, perché non avete apposto la fiducia e vi siete messi d'accordo. Adesso vedremo anche se la Lega ritirerà le proprie firme per i voti segreti. Qua dentro vedremo un sacco di cose. D'ANNA *(ALA-SCCLP)*. Ci sapete dire quale dei diritti costituzionali è maggiore? Il diritto all'istruzione o il diritto alla salute? ai bambini non vaccinati negherete il diritto all'istruzione. Mi sapete dire qual è quello prioritario in questo Stato etico? Quale di questi due diritti è maggiore? Non lo sapete, perché state ponendo in essere una volgare prova di forza. State dando la peggiore dimostrazione della politica politicante. Altro che grandi tematiche e grandi idealità. un giorno vedremo che si tratterà solo di sordidi interessi. Signor Presidente, nella mia breve carriera politica, tra la montagna dei dubbi e la montagna delle certezze ho sempre preferito scalare la montagna dei dubbi. modo abbiamo chiesto che si aprisse questo dibattito in Parlamento, visto che nel Paese si è aperto un dibattito straordinario su questo argomento, proprio perché sono tantissimi i dubbi che nutriamo rispetto alle certezze che qualcuno evocava anche negli interventi che mi hanno preceduto. Mi sono anche peritato (non so quanti dei miei colleghi lo abbiano fatto) di incontrare chi in piazza ha manifestato. Caro senatore D'Anna, ho incontrato per un'ora e mezza coloro che oggi erano in piazza. C'era una delegazione, è venuta a trovarmi e mi sono confrontato con loro. È stato importante e interessante, perché hanno offerto tanti punti di vista: tanti convincimenti definitivi sul fatto che non si dovesse vaccinare, vaccinare, altri che invece sostenevano che non si dovesse inserire l'obbligatorietà del vaccino, mentre altri contestavano i numeri che il Ministro ha evocato anche prima nel suo intervento. Quindi, vi è un dibattito franco, aperto e importante.

continuare questo percorso. Abbiamo davanti un percorso di circa 300 emendamenti. Ho la sensazione, perché abbiamo anche noi parlato con il Governo, che ci sia la possibilità di migliorare fortemente il provvedimento uscito dalla Commissione. questo do atto, ma lo vedremo nei fatti e negli emendamenti che saranno messi in votazione, se questo avverrà veramente e mi auguro che accada. Ci sono le condizioni, da un lato, di rispettare

è contro i vaccini. Siamo per i vaccini che sono utili e che potrebbero essere utili per i nostri figli. La dichiarazione che il Governo non aveva titolo per fare un decreto-legge non è mia, ma di un signor che porta il nome di Ferdinando Imposimato.

Ci siamo interrogati - e lo chiedo a lei, signor Presidente del Senato perché in lei confido - se quello che c'è scritto nei giornali e quello che si sente oggi corrisponde alla realtà oppure no. Il ministro Lorenzin - che non entra nel merito della discussione perché la riconosco come Ministro ma credo che, sotto il profilo sanitario, abbia le competenze perché qualcun altro gliele ha consegnate, ma lei personalmente non le ha

È vero o no che a fare questo piano sono state due persone di cui una ha usufruito indirettamente della sponsorizzazione per una cattedra universitaria e porta il nome di Ricciardi? È vero o no che c'è un personaggio che porta il nome di Pecorelli che nel 2015 è stato messo alla porta perché aveva dei rapporti non chiari e conseguentemente c'era conflitto di interesse? *(Ilarità)*. È vero o no che chi ha partecipato alla costruzione di tutto questo percorso sono quattro multinazionali e due multinazionali hanno sponsorizzato con con 600.000 euro la cattedra di un professore universitario e l'associazione legata a questo professore è fatta di figli, nipoti e cugini?

Quando c'è una perplessità, noi abbiamo l'obbligo di fermarci, chiarire e poi andare avanti. Chi vuole andare avanti a ogni costo è complice e compromesso e mi sento di dirlo davanti agli uomini e davanti a Dio. Signor Presidente,

in coerenza con l'intervento che ho svolto questa mattina in discussione generale e rafforzato in questo convincimento anche dall'intervento del ministro Lorenzin, annuncio in dissenso dal mio Gruppo il mio voto contrario sulla proposta di non passare

con una valutazione che vorrebbe recuperare il senso di una dialettica matura e responsabile. Noi siamo nell'Aula del Senato il confronto e il dibattito che vi si svolge dovrebbe agevolare, favorire e promuovere la migliore comprensione degli argomenti, allontanando lo spettro dei nodi ideologici che sembrano addensarsi attorno ai temi delicatissimi di cui stiamo parlando e a cui ci dobbiamo accostare privi di pregiudizi e soprattutto, se mi è permesso, documentando in modo responsabile e corretto le dichiarazioni che si fanno. Sugli inquinanti presenti nei vaccini, finanche le numerosissime analisi commissionate dai movimenti anti-vax hanno certificato che la presenza di mercurio è talmente

cui, per un verso, abbiamo assistito alle tendopoli di chi ha sostenuto, promosso e spinto il legislatore a consentire l'accesso a metodiche terapeutiche prive e, dall'altro, laddove il fondamento scientifico esiste (poiché è acquisito a livello internazionale che le pratiche vaccinali rappresentano la più grande conquista dopo la potabilizzazione dell'acqua) abbiamo introdotto, su basi assolutamente gravi di insinuazioni e di infondatezza scientifica clamorosa, la cultura del sospetto che induce la popolazione, non a essere contraria, ma ad essere confusa.

quei coni d'ombra che ancora esistono, per consegnare al Paese non solo la verità, ma anche un provvedimento che tuteli realmente la salute della gente.

del percorso che il Ministro della salute ha indicato circa l'obbligatorietà dei vaccini. Ne siamo convinti, perché ci sentiamo la responsabilità della collettività, ci sentiamo la responsabilità di uno Stato che di fronte ai bambini, che sono certamente i più indifesi, ha la necessità di garantire loro una copertura vaccinale importante. Noi, signor Presidente, siamo pronti a discutere emendamento su emendamento in quest'Aula, forti di questa convinzione e con il coraggio di sapere che stiamo facendo una cosa importante per la nostra Nazione. Adesso e anche nelle prossime legislature noi continueremo a perorare questa necessità, questa copertura vaccinale che negli anni si è assolutamente abbassata. Signor Presidente, siamo anche abbastanza preoccupati di quello che abbiamo sentito in quest'Aula nel corso di questo dibattito; e lo voglio dire in maniera molto serena. agli amici della Lega del Veneto, che sostengono che attraverso il convincimento, la comunicazione, il rapporto, il dialogo e la non obbligatorietà sono riusciti comunque ad avere buone coperture vaccinali, noi sommessamente vogliamo ricordare i dati che in quest'Aula e nella Commissione sanità abbiamo sentito, anche

abbondantemente sotto il 90 per cento, e noi sappiamo bene che l'Organizzazione mondiale della sanità richiede una copertura di almeno il 95 per cento per avere quell'effetto gregge di copertura e di sanità su tutto il nostro territorio nazionale. E ancora, signor Presidente, io vorrò rileggermi con molta attenzione le dichiarazioni che ultimamente ha fatto il senatore Scilipoti Isgro', il quale compromesso e complicità. Voglio capire bene come ha agganciato questi concetti, perché forse sono stata poco attenta. Voglio rileggere quelle parole, che sono veramente scandalose in un'Aula così seria, che sta trattando seriamente un tema del genere. *(Applausi dai come ha legato questo essere complici rispetto a tutto il dibattito che c'è fuori, un dibattito che certamente è confuso e che noi rischiamo, con queste dichiarazioni, di rendere ancora più confuso. E infine voglio dire una cosa al senatore Paolo Romani, che è una persona estremamente seria. Noi apprezziamo molto quello che egli ha detto e apprezziamo il fatto che voglia misurarsi sugli emendamenti, per migliorare questo provvedimento. Ma, senatore Romani, non è che si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Siate responsabili anche voi sugli emendamenti che da questo punto di vista sono contro il

Signor Presidente, devo dire che non mi sarei aspettato, dopo lunghe discussioni in Commissione, che arrivassimo in Aula così divisi e così arrabbiati.

cercare di convincere le persone che non c'è un grosso pericolo, se non una supposta epidemia di morbillo.

Quanti morti ha provocato? Centinaia di morti, come lei dice? Non mi risulta e non risulta a nessuno. Detto ciò, io sono perfettamente convinto dell'importanza dei vaccini; so perfettamente, avendo studiato su libri di medicina e non su altri libri, che, dopo la potabilizzazione dell'acqua, la vaccinazione è stata la più grande scoperta, per risolvere a livello mondiale problemi di sanità. Però questo ora non vale più nei Paesi evoluti; vale molto per i Paesi del Terzo mondo. Noi abbiamo altre epidemie gravi, che ho cercato di farvi capire anche nel mio intervento. Le nostre epidemie si chiamano diabete, ipertensione,

diversi discorsi e ho ascoltato anche l'intervento del senatore D'Anna; devo dire che alcune cose che ha detto sono estremamente condivisibili, senatore D'Anna. una cosa però che mi preoccupa: perché, visto che in Commissione molti di questi emendamenti che noi stiamo discutendo sono passati con undici voti contro dieci, lei non è mai venuto in Commissione a riferirci le sue idee? Perché alcuni si sono allontanati dalla Commissione quando potevamo discutere di queste cose? Questa mattina ho fatto un intervento critico su questo modo di portare avanti l'obbligatorietà vaccinale. Molte di quelle persone che sono fuori a protestare, protestano non contro le vaccinazioni, ma contro il metodo, contro la maniera in cui vengono impostate, contro l'impossibilità di fare una vaccinazione singola,

Perché io che ho tempo, ho molto tempo per parlare con i pazienti, spiego loro perché ci si può vaccinare più tardi, cosa che molti medici non fanno per mancanza di tempo. Se noi rompiamo, come ho detto questa mattina, questo rapporto di fiducia che abbiamo stipulato con i nostri pazienti, se un paziente mi si mette davanti e mi dice: «lei è costretto a dirmi che devo fare i vaccini altrimenti la radiano»,

Se un Ministro o qualcuno di noi dice delle grosse bugie e delle grosse sciocchezze, poi non siamo più credibili: è questa la differenza fondamentale; è questo su cui dobbiamo lavorare. Ho anche detto che, siccome ritengo che i cittadini devono capire che lo Stato è dalla loro parte e non contro di loro, non voglio sentir parlare di complottismo,

scientifico. Sono favorevole al non passaggio agli articoli, per un solo motivo: spero che tutti coloro che hanno sbraitato qui dentro contro questi emendamenti e fanno parte della Commissione sanità,

abbiamo apprezzato tutti il lavoro della Commissione. Se tornare in Commissione sanità serve per vedere le facce di coloro che non ce l'hanno messa, sono convinto che questo sia un passaggio utile.

e vorrei motivare la ragione. Prima, però, chiederei ai colleghi che hanno insinuato un'eventuale interesse personale di coloro che sono a favore di questo provvedimento, di ritirare questa affermazione perché è inaccettabile. È inaccettabile in particolare nei confronti di coloro, come il sottoscritto, che tutti i giorni sono in competizione con le multinazionali e sanno perfettamente qual è la loro azione prevaricatrice nel nostro Paese. Chiederei altrettanto posizionamento quando si discute di altre questioni sulle multinazionali, caro collega D'Anna.

del nostro mercato a una concorrenza vera. Vedremo cosa farete quando esamineremo il provvedimento sulla concorrenza. Resto però sul merito, colleghi. Romano - che in Svezia non c'è l'obbligatorietà per legge della vaccinazione, ma in Svezia non ci sono neanche i cartelli «Qui si buttano rifiuti lungo le strade». Cari colleghi, noi abbiamo bisogno dell'obbligo della vaccinazione, perché il nostro Paese è molto disponibile a inseguire le "farlucche", come sta accadendo con questo provvedimento. Qui non c'è bisogno di dimostrare niente; c'è bisogno di prendere atto di cinquant'anni di storia della sanità del nostro Paese, di quali sono state le conquiste nel nostro Paese. E se oggi non c'è un pericolo imminente è perché ci sono state quelle conquiste, quell'azione obbligatoria, quel contributo dello Stato alle classi più povere di questo Paese che avevano bisogno Vi siete dimenticati di questo. Non nel 1948, nel 1950, nel 1960 e in tanti altri anni ancora. Dico allora questo, cari colleghi: la scienza ci dimostra che i vaccini non fanno male: fanno bene, ci mettono al riparo. Quando ci saranno proposte più avanzate, le esamineremo con grande apertura culturale, scientifica, mentale, etica, religiosa, politica, mettetela come volete. Oggi la vaccinazione è lo stadio più avanzato di prevenzione per tutta una serie di malattie, in una situazione anche di grande passaggio, di rapidità di persone da un mondo all'altro, che si portano dietro fattori positivi ma anche vecchi e nuovi rischi. Quindi, io sono del parere, caro Ministro, che dobbiamo mettere il cartello: «Qui la vaccinazione è obbligatoria». Quando non ce ne sarà più bisogno, toglieremo anche i cartelli dalle strade che dicono di non buttare l'immondizia lungo la strada, ma io che giro l'Italia ne vedo troppa e ne vedo troppa proprio dalle parti dove queste voci si sollevano con grande indignazione.

dell'idea che occorra intervenire nel merito degli emendamenti e provare possibilmente a migliorare il provvedimento. Mi preme anche sottolineare certi confronti che sono stati fatti, perché, come non si possono confrontare le mele con le pere, non si può confrontare una reazione avversa di un caso

l'obbligo di vaccinazione nei vari Paesi senza tenere presenti le condizioni precise di ciascun Paese. Sottolineo anche che le cose non sono come sono state dette, perché in 14 Paesi europei vige l'obbligo anche un numero superiore a sei vaccinazioni. Da ultimo, alla senatrice Bianconi vorrei dire che questa non è una Repubblica presidenziale, ma neanche una Repubblica senatoriale: è il Parlamento che decide insieme quali sono gli emendamenti che rendono un provvedimento migliore o no.

ad avere grandi aberrazioni. Chi si deve occupare di una materia se non uno che ha avuto a che fare con essa, nel senso che ha studiato, ha le competenze, ha approfondito e per cui magari ha

né delle case farmaceutiche per fare un percorso di carriera, che magari suscita le gelosie di qualcun altro che vorrebbe stare al posto suo o magari al posto della Ministra della salute. Succede così, purtroppo nella vita non tutti possono avere quello che vorrebbero. Quindi, a questo punto non posso chiamare il giardiniere o il fruttivendolo sotto casa, che di sicuro non hanno mai avuto a che fare con una casa farmaceutica, uno studio o una rivista

la persona giusta che mi aiuta a fare un provvedimento, perché di vaccinazioni non ne saprà nulla. Usciamo da questi schemi, perché queste sono rigidità che ci impediscono di vedere ciò che è palese è palese se semplicemente sgombriamo la mente da certe ideologie e da certi pregiudizi e cerchiamo, invece, di migliorare nel merito il provvedimento. Ne abbiamo occasione, perché consideriamo che, purtroppo, con tutti gli errori che sono stati fatti nella gestione di questo provvedimento, non andare avanti oggi significherebbe avallare tutte le *fake news*, tutto il complottismo che ha portato a un obbligo che potevamo evitare con maggiore responsabilità da parte di tutti, anche e soprattutto di tanti medici.

hanno altri interessi. Dico solo una cosa e concludo. I vaccini devono essere puliti: vaccini anche con piccolissime quantità di mercurio o di allumino non devono esserci. Vanno dati vaccini puliti. Se si può fare, lo si deve fare. Chi non lo fa, si assume la responsabilità morale ed etica di eventuali reazioni avverse e di morti che sicuramente ci saranno: sta a voi e alla vostra coscienza.

fermi! Vagliamo tutto. Non può dividere: si rende conto che sta dividendo una Nazione? È questo che vuole? Si fermi, faccia vagliare, prendiamo tempo: solo questo le chiedo.

3.34, 3.47 e 5.15 in quanto estranei al contenuto del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Risultano altresì inammissibili gli emendamenti 1.12 e 1.13, che recano una delega legislativa in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione, nonché le proposte 1.16 e 1.17, in quanto delegano ad un decreto ministeriale l'individuazione delle vaccinazioni obbligatorie, in contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. In relazione ai subemendamenti presentati, la Presidenza dichiara inammissibili le proposte 1.98 (testo 2)/1, 1.127/1, 1.127/2, 1.127/4, 3.9/1, 3.9/2,

e nella miglior maniera garantiti e controllati da parte dello Stato. Al comma 3 si stabilisce pertanto che «Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini di cui al presente articolo è affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare con sede a Firenze». anche a fugare tutte le paure esistenti, motivate o meno. Noi riteniamo che molte siano motivate, considerando qual è stata la classe politica e quali gli scandali che hanno costellato il panorama delle scelte relative ai farmaci e a chi doveva fornire cosa.

se da zero casi si passa a un caso, per lui c'è un aumento del 100 per cento e, quindi, siamo in epidemia. Questo è l'Istituto superiore di sanità al quale abbiamo affidato la

il provvedimento non deve essere assolutamente coercitivo. Il secondo emendamento è l'1.76, con il quale chiediamo che, successivamente alle vaccinazioni,

quarto emendamento che illustro, al quale invito i colleghi a prestare attenzione, è l'1.91. Faccio qui riferimento anche a quello che ha detto prima il senatore Bianco sugli esoneri dell'obbligo della vaccinazione. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'articolo 1 prevede che, per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, vi sia l'esonero dell'obbligo della relativa vaccinazione. vaccinazione. Ebbene, noi vogliamo integrare questo comma dicendo che non può essere somministrato all'individuo che ha l'immunizzazione per avvenuta

propone una mediazione sulla obbligatorietà dei vaccini. La nostra proposta (non solo nostra, ma anche di altri) è quella di mantenere l'obbligatorietà dei quattro storici vaccini obbligatori, più quello sul morbillo, sul quale vi è una reale preoccupazione. sono poi degli emendamenti che propongono la vaccinazione degli operatori sanitari, sui quali già questa mattina ho detto che vi era un problema di copertura. Ho invitato però il Governo (e penso si stia lavorando in questo senso)

Prego,

2)/1 è stato dichiarato inammissibile.

parere contrario

premettere il seguente periodo: "In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 4 le parole "in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui al comma 1"».

ritiro dell'emendamento 1.115, perché si ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 1.116, che segue. Quindi un invito al ritiro o un parere favorevole, ma è preferibile la formulazione successiva.

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, possono autorizzare la somministrazione da parte dei medici che hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari dei vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per l'attuazione di cui al comma 1 anche in ordine ai profili relativi alla certificazione dell'avvenuta vaccinazione».

e propongo la trasformazione in ordine del giorno

per quanto mi consta, il Governo si era impegnato a trovare la copertura; quindi, pensiamo che il parere debba essere favorevole perché riteniamo che il Governo abbia trovato la copertura. Su questo punto vorremmo avere una certezza.

Certo, Centinaio, abbiamo ragione a migliorare un provvedimento. Abbiamo proprio ragione e continuiamo a cercare di migliorarlo.

era un parere favorevole del relatore.

che riguardava la vaccinazione degli operatori sanitari, riteniamo che debba essere un emendamento e non un ordine del giorno e anche su questo argomento chiedo il parere del Governo.

alle necessarie verifiche. Per quanto attiene la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, non avendo ancora ricevuto un testo, ho tenuto una posizione cautelativa: se vi è un testo su cui c'è accordo tra tutti, per me va bene.

ed ero d'accordo con l'idea di un accantonamento per un approfondimento, perché dai pareri che avevamo ricevuto in precedenza della Commissione bilancio non avevamo riscontrato nulla di ostativo.

finestra"). Sulla riformulazione dell'emendamento vorremmo qualche chiarimento, per capire qual è la riformulazione e qual è l'emendamento,

ai sensi dell'articolo 81, di trasformarlo in ordine del giorno. Il Governo, che si è testé pronunciato, ha ribadito la conformità al parere del relatore.

Signor Presidente, capisco che sia tutto molto complicato e prego i colleghi di avere un po' di considerazione, perché non è semplice lavorare in queste condizioni. Abbiamo

rilevo un procedimento piuttosto anomalo e al limite dell'accettabilità, per cui un singolo senatore, per quanto Capogruppo, chiede al Governo di rivedere il proprio parere, sulla base di un'informazione extraparlamentare, di cui evidentemente gode e di

Presidente, ove

non essendomi sufficientemente chiara la motivazione e volendo anche avere il tempo di acquisire la relazione tecnica,

Presidente, la tranquillizzo, non ho niente da accantonare.

dal farlo, perché vengo da una militanza politica e so che gli accordi tra forze politiche

non basta scrivere «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» per bypassare il giudizio della Commissione

non sto ponendo il voto di fiducia, ma sto cercando di introdurre una parola di rasserenamento nella discussione. Signor

qui stiamo ragionando di emendamenti che, originariamente, erano della Commissione. Così è per l'emendamento 1.1500 che ha raccolto, evidentemente, essendo un emendamento della Commissione, il sentire di una gran parte della Commissione medesima rispetto a un indirizzo, quello della vaccinazione di tutti gli operatori sanitari e scolastici, che risponde a una esigenza di razionalità, che io ben capisco possa essere stata condivisa da colleghi di diversi Gruppi parlamentari.

Quindi, le due questioni sulle quali la Commissione bilancio ha dovuto - e giustamente, perché non vi è una norma di copertura finanziaria né è prevista la spesa del minor gettito ai sensi dell'articolo 81 riguardano due emendamenti che non appartengono a una parte politica piuttosto che all'altra, ma sono il frutto di una valutazione che è stata talmente larga da far diventare questi emendamenti della Commissione. Dopodiché, ovviamente, i colleghi possono avanzare la legittima richiesta di rivisitazione delle valutazioni circa l'articolo 81, ma con la stessa identica fortuna, in assenza di una

ovviamente, non significa che a queste esigenze non si possa rispondere altrimenti. E mi riferisco non soltanto allo strumento dell'ordine del giorno, che pure ha una sua piena e compiuta legittimità, ma anche al fatto che alcune di queste questioni, come per esempio quella riguardante la vaccinazione obbligatoria di minori non accompagnati, sono di fatto risolte. L'approfondimento che abbiamo condotto questa mattina insieme alla Ministra

Senatore Gaetti, le dico quello che a me risulta per un approfondimento al quale ho assistito personalmente e la prego di non dubitare della mia buona fede. Non vengo mai a raccontare in Aula cose delle quali non sono personalmente consapevole. E questo per mia misura di vita.

e le questioni finanziarie sono serie e riguardano temi trattati e accolti dalla Commissione. Per quanto mi riguarda - ma la responsabilità politica del provvedimento non è mia - sarà fatto tutto il possibile per venire incontro a esigenze condivise e che non possono allo stato essere assistite da copertura finanziaria e, quindi, da un parere favorevole *ex* articolo 81

gli italiani, attraverso gli sms solidali, hanno donato qualcosa come 32 milioni di euro. Di questi 32 milioni, 17,5 sono toccati, nella ripartizione, alla Regione Marche. Oggi, alcuni mezzi di informazione hanno reso note le volontà della Regione Marche di come destinare le risorse che i cittadini generosi hanno donato.

e addirittura, per il recupero della grotta sudatoria di Acquasanta Terme, verranno utilizzati 3 milioni di euro. Credo che la Regione Marche sia letteralmente impazzita. Si tratta di risorse che i cittadini avevano donato, in occasione del terremoto, per far fronte alle prime necessità e per mettere gli enti pubblici nella condizione di superare una calamità che è stata davvero drammatica. Non si può pensare che tali risorse possano essere utilizzate in maniera così impropria. impropria. Non credo che in Italia vi sia un solo cittadino che dona due euro in occasione di una calamità per far costruire una pista ciclabile oppure per mettere in sicurezza una grotta come quella sudatoria del Comune di Acquasanta Terme.